di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali*** *(Approvato dalla Camera dei

L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Belisario e da altri senatori, concernenti il sottosegretario Nicola Cosentino. Ciascun Gruppo avrà a disposizione 18 minuti, comprensivi delle illustrazioni, degli interventi in discussione e in dichiarazione di voto.

di essere il più possibile sintetico ed attinente al tema. C'è un famoso romanzo, che molti in quest'Aula hanno sicuramente letto e che, con ogni probabilità, converrebbe rileggere. È un romanzo di Sciascia, che si intitola «Il contesto»; un romanzo molto bello, che ci dà un'indicazione su come affrontare questa vicenda, su come porci rispetto a tale questione e sul metodo che dobbiamo adottare. Il metodo è, in primo luogo e per l'appunto, quello di individuare il contesto in cui la vicenda si colloca.

La mozione n. 43 è molto semplice: impropriamente ed atecnicamente, essa è stata indicata come mozione di sfiducia individuale nei confronti del sottosegretario Cosentino. Ricordo che esiste la possibilità di mozioni di sfiducia individuali, ma esse riguardano soltanto i Ministri della Repubblica e non già i Sottosegretari. L'oggetto di questa mozione è molto semplice e riguarda l'opportunità che il Governo della Repubblica inviti il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino a rassegnare le dimissioni; ciò in relazione al suo coinvolgimento, nella qualità di indagato per reati gravi, in un'indagine della procura della Repubblica e della DIA di Napoli. Il contesto di cui dicevo è palese, per molti aspetti evidente e davanti a tutti; ogni giorno esso si arricchisce di nuovi tasselli. Non alludo all'ordinanza di applicazione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare, arrivata molto tempo dopo la proposizione della nostra mozione, ma alludo, ad esempio, ad una notizia di oggi, che leggiamo sui giornali e sulle agenzie e di cui darò una sintesi. 120 milioni di euro, 2 dei quali in contanti, è il valore dei beni sequestrati dalla DIA di Napoli a carico di persone ritenute riciclatori per conto del clan dei casalesi. L'operazione, detta "Faraone", in particolare ha individuato soggetti vicini al clan che, per riciclare denaro, acquistavano proprietà in aste giudiziarie (vi prego di ricordare il concetto dell'asta giudiziaria, che ci servirà fra poco),

del membro del Governo di cui oggi ci occupiamo? Sempre in merito al contesto, in quest'Aula, pochi giorni fa, è stata approvata una norma che ha suscitato e suscita dure polemiche, sulle quali non voglio tornare. però rileggere tale norma, che riguarda la possibilità di procedere alla vendita di beni confiscati alle organizzazioni criminali: «Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*» - i beni in discorso - «e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, il dirigente del competente ufficio del territorio... Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, ...da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata». Lasciatemi fare una domanda provocatoria: ove il sottosegretario Cosentino volesse acquistare uno dei beni confiscati alla criminalità organizzata, magari proprio uno di quelli sequestrati nell'odierna operazione, chiedo ai membri del Governo, chiedo agli appartenenti alla maggioranza e in particolare a chi più di altri è attento ai temi del contrasto al crimine, gli appartenenti al partito della Lega, potrebbe farlo? Cosa dovrebbe dire il prefetto, dipendente del Governo cui il sottosegretario Cosentino appartiene? Dovrebbe dire che si tratta di soggetto riconducibile alla criminalità organizzata? Cosa dovrebbe fare il dirigente dell'Agenzia del demanio? Che parere dovrebbe esprimere il Commissario straordinario? Mi piacerebbe, nel corso del dibattito che seguirà questa breve illustrazione, sentire l'opinione degli appartenenti alla maggioranza su questa semplice domanda: potrebbe il sottosegretario Cosentino acquistare i beni oggi sequestrati un giorno che fossero confiscati? Se la risposta fosse negativa, come potrebbe il soggetto che non sarebbe per la legge da voi stessi approvata una settimana fa abilitato ad acquistare quei beni fare il Sottosegretario all'economia e alle finanze (dico solo per inciso, il Ministero da cui dipende la Guardia di finanza)? Noi non possiamo e non vogliamo sostituirci all'autorità giudiziaria per esprimere giudizi di colpevolezza, ma non possiamo e non vogliamo - e nemmeno voi potete farlo - sostituirci all'autorità giudiziaria per esprimere giudizi di innocenza. La chiave di volta, la soluzione di questa vicenda è contenuta, come per molte altre vicende, nella Costituzione, all'articolo 54, in quella norma che dice: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Disciplina e onore che fanno riferimento ad una categoria concettuale, una funzione che non è una proprietà privata del soggetto investito ma qualcosa che si fa nell'interesse della collettività e che bisogna essere capaci di abbandonare nel momento in cui la permanenza in quella posizione sia lesiva dell'onore individuale e dell'onore delle istituzioni. L'onore è anche saper fare un passo indietro, collettivo e individuale. Concludo con una citazione da un grande scrittore, Anton Cechov, che diceva che l'onore non si può togliere, si può solo perdere.

di cui sono componente, si è recata a Caserta, il dato che più impressionò tutti i

fu la considerazione espressa dai vertici delle articolazioni statuali - dal prefetto, al questore, al comandante dei carabinieri - sul fatto che in quei luoghi era persa la possibilità di individuare con nettezza la linea di confine tra il malaffare e la legalità. Diversamente che in altri territori, lo Stato comunicava al Parlamento questa grande confusione che investiva la collettività del casertano. casertano. Ognuno di noi si sentiva portatore di un'esigenza, sentiva la necessità che lo Stato, in quei territori dove la linea di confine tra malaffare e legalità si è persa, fosse in grado di dimostrare la sua autorevolezza e la sua concreta espressione, anche attraverso gesti che potessero significare una scelta ben precisa in direzione della legalità e per sconfiggere il malaffare. Oggi, da un'intervista resa dal senatore Quagliariello ad un quotidiano, apprendiamo che sulla vicenda della quale ci stiamo occupando entra in gioco il problema ed il profilo dello Stato di diritto. diritto. Il senatore Quagliariello, cioè, spiega cosa significhi difendere lo Stato di diritto. Egli dice: «Solo così è possibile capire cosa fare per difendere lo Stato di diritto. E oggi, per salvaguardare l'autonomia della politica rispetto alla magistratura ed ai pentiti, è necessario che il passo indietro non ci sia». sia». È necessario, cioè, per difendere lo Stato di diritto, che il sottosegretario Cosentino, indagato per concorso esterno in associazione camorristica, del quale è stata chiesta la misura cautelare in carcere, rimanga intonso dai giudizi che la politica deve esprimere nel nome dello Stato di diritto in quanto lo Stato di diritto, evocato dal senatore Quagliariello, si contrappone alla magistratura ed ai pentiti. La magistratura, cioè, diventa il soggetto antagonista dello Stato di diritto. A noi provoca sicuramente un giudizio di non condivisione di siffatta impostazione.

Per fare ciò ci sarà la magistratura. Noi stiamo soltanto sollevando un problema di competenza dell'Assemblea sovrana: nel nome dello Stato, esiste un profilo di opportunità, laddove un componente del Governo raggiunto da gravi accuse valutate in questa prima fase dalla magistratura che attraverso la sua valutazione è giunta alla conclusione di chiederne l'arresto? Esiste

tra legalità e malaffare, che è presente anche valutando la trasparenza dei componenti del suo Esecutivo? Nell'ambito delle opportunità, e quindi delle valutazioni che afferiscono alla politica - ma la politica non può non farsi carico di questa esigenza può veramente assumersi che non sussista una ragione di opportunità? Noi non vogliamo pronunciare giudizi; vogliamo che lo Stato possa presentarsi ai cittadini con la veste di chi può con trasparenza guardare negli occhi i cittadini onesti, quei cittadini onesti che vogliono dallo Stato un segnale, il segnale che noi vorremmo inviare e che è diverso da quello auspicato dal senatore Quagliariello, che invece raggiungerebbe le organizzazioni criminali come segnale di debolezza. alla sovranità di quest'Assemblea di valutare politicamente le ragioni di opportunità e quindi di sollevare il problema al Governo, per cui nel nome dell'opportunità debba avviare la procedura di revoca dell'incarico governativo conferito al sottosegretario Cosentino.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi nella riunione della Commissione antimafia, della quale mi onoro di far parte, abbiamo avuto un'audizione con il ministro dell'interno Roberto Maroni,

casi di particolare successo in questo senso, che riguardano proprio Caserta, proprio la Campania.

avviate indagini e commissioni di accesso per arrivare allo scioglimento dei Comuni nei quali c'è il sospetto che ci sia l'infiltrazione della camorra.

in cui ancora siede un sottosegretario, l'onorevole Cosentino, sul quale pesano gravi sospetti e per il quale c'è stata anche una richiesta di arresto. Io non voglio citare questioni giuridiche e neanche giudiziarie; non voglio neanche pensare che qui si possa trattare di queste. Vorrei parlare di etica nella politica;

che, sfiorati da sospetti, non hanno esitato che pochi minuti prima di prendere la decisione - una scelta etica, di trasparenza - e lasciare quelle istituzioni che devono essere al di sopra, esse sì, di ogni sospetto, perché sia intonso il prestigio e la dignità dei luoghi nei quali la politica c'è. Pertanto chiediamo una riflessione in questo senso e perciò chiediamo le dimissioni. È vero, si è innocenti fino a prova contraria, e questo vale per tutti i cittadini, ma, mi chiedo, se in una scuola vi fosse una maestra accusata di lucrare i soldi delle gite scolastiche noi, con coscienza tranquilla, vi lasceremmo i nostri bambini? una nuova finestra"). Sono presenti in tribuna gli studenti del Liceo scientifico «Enrico Medi» di Montegiorgio, in provincia di Ascoli Piceno. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, nell'Italia borbonica spadroneggiavano i pentiti: li si definivano testimoni di Stato e questo bastò più di un secolo fa a far pronunciare a Gladstone nel Parlamento inglese il famoso discorso sulla negazione di Dio elevata a sistema politico. Parole forti, ma nella storia patria quel discorso di Gladstone fu per Cavour, Mazzini e Vittorio Emanuele importantissimo, forse decisivo. Sicché oggi la prospettiva di tornare ai testimoni di Stato non ci entusiasma e dovrebbe preoccuparci: i pentiti dichiarano, il giornalismo cosiddetto investigativo ne riproduce i verbali, le procure molto spesso lo consentono, nessuno controlla e verifica un bel niente: l'Italia borbonica sembra resuscitata. Al nostro esame c'è il lungo e faticoso sentiero di un giovane parlamentare della provincia di Caserta, al quale accadde di conquistarsi stima e apprezzamento, non facili, di un uomo del profondo Nord, Giulio Tremonti.

recepito in pieno e senza verifiche, il muro delle dichiarazioni dei pentiti, delle violazioni del segreto di indagine e delle menzogne più turpi che pretendono di farsi verità rivelate e rivelatrici. Con qualche eleganza il senatore Carofiglio ha citato "Il contesto" di Sciascia; con un linguaggio un po' più crudo, nella mozione Zanda, al penultimo capoverso, si definiscono "gravi delitti, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi", quelli che al momento, me lo consenta l'amico Zanda, sono soltanto ipotesi e congetture, su cui tra l'altro non è il Senato che deve pronunciarsi. E poi, considerazione non marginale, la nostra Costituzione non prevede in nessuno dei suoi commi e articoli che tocchi all'imputato dimostrare pienamente - come si dice nella vostra mozione - la sua piena innocenza. ferma restando la libertà di esprimersi anche con linguaggio più crudo, non vorrei che il Parlamento cedesse all'acquiescenza, a mio giudizio esagerata, nei confronti del giornalismo investigativo. Anche con l'elegante richiamo di collegialità si richiama la legge sulla Presidenza del Consiglio, la n. 400 del 1988), sarebbe nei fatti la parola dei camorristi a far dimettere dall'Esecutivo il sottosegretario Cosentino. Egli, voi dite, ormai ha solo il diritto di pensare a difendersi, ma questo diritto non può essere messo fra parentesi, perché la sua difesa non dovrebbe esplicarsi nel processo invece che dal processo, come altre volte si amava dire, perché per lui il processo non c'è: solo dimissioni e arresto. Quanto al dibattimento, vario ed eventuale, esso è al momento assorbito nelle indagini. Questo è allora il punto. Credo che in buona fede, l'amico senatore Li Gotti, polemizzando con Gaetano Quagliariello, abbia in realtà rievocato le parole che disse il senatore Giovanni Pellegrino.

siamo ai limiti dello Stato di diritto e della Costituzione; non vorrei che venisse un giorno in cui saremo anche fuori del diritto alla giurisdizione». Si tratta di quell'articolo della Costituzione citato dal collega Li Gotti. Allora, se non vogliamo risalire a precedenti dell'Italia borbonica, dobbiamo guardare con più onestà anche al giornalismo investigativo,

né marginale né nasce da cavillosità e credo che il senatore Zanda possa darmene atto, perché è molto amaro che dal presupposto ‑ falso di un ruolo di Cosentino al CIPE si sia approdati al passo successivo, non meno falso, di una piovra camorrista insediatasi al CIPE del resto, nello stesso errore, con la stessa buona fede di Zanda e degli altri, la scorsa settimana è incappato anche il neoparlamentare europeo De Magistris: eravamo nello studio televisivo

camorra, che su Cosentino - lo dicono le mozioni - incomberebbe da tantissimi anni, quasi da quando lo conosco, e con la quale egli finora ha cercato di convivere con la mitezza e l'ironia, ma anche con la sincera sofferenza delle persone perbene. Gli capitò una volta di chiamarla il suo angelo custode invisibile, scherzandoci sopra, ma con una compostezza che era l'altra faccia della medaglia. Su di lui, del resto, nelle vostre mozioni dite che s'indaga da più di tre lustri, più di 15 anni, ma sempre in modo sleale, senza alcun rispetto di quel codice dei galantuomini che dovrebbe essere - parole di Piero Calamandrei - il codice di procedura penale (ma ovviamente per Calamandrei il codice penale era il codice dei mariuoli). E allora, colleghi, dopo più di tre lustri, del suo diritto ad un giusto processo - magari nei modi, nei tempi e nelle forme dell'articolo 111 della nostra Costituzione - non c'è alcuna traccia: non c'è nelle pagine de «L'Espresso» (forse bisognava aspettarselo), ma non c'è neanche nella recente richiesta per lui di misura cautelare custodiale. Proviamo, colleghi, a non ragionare esclusivamente in termini di questioni *ad personam*; almeno per una volta, per rispetto a quella modica quantità di *human rights* a cui avrà diritto anche il sottosegretario Cosentino. Proprio le premesse richiamate nelle mozioni qui illustrate implicano una considerazione diversa. Le indagini - benissimo - abbiano il loro ambito e il loro spazio, ma senza le furbizie e i giochetti (fra il nascondino e il ping pong) delle iscrizioni varie ed eventuali nel registro delle notizie di reato, senza che sui verbali dei pentiti pascolino giornalisti cosiddetti investigativi. Altro che pratiche a tutela al CSM: la vera tutela e garanzia della magistratura italiana dovrebbe essere cancellare il concorso esterno! Quello che la procura di Napoli si concesse a suo tempo contro Enzo Tortora fu grave (non dico che fu infame perché non è il mio linguaggio), e non deve ripetersi. Lo ha detto un deputato radicale, l'onorevole Turco, evidentemente legato ancora alla tradizione di Calamandrei, e questo gli fa onore, non meno del suo dissenso politico dalle posizioni mie o di altri. I tempi di un procedimento non possono restare tra le varie ed eventuali della lotta politica:

a proposito della durata delle fasi del processo, credo che non si possa continuare ad evocare in modo così tendenzioso la questione di costituzionalità e/o di incostituzionalità. Non entro nel merito

che qualcosa di una concezione liberale della procedura penale ci ha detto in quell'occasione. Per noi del PdL i valori costituzionali hanno priorità diverse dalle vostre, ad esempio la difesa dell'individuo da una persecuzione giudiziaria, da un'azione penale che possa essere persecuzione giudiziaria protratta nel tempo. È un diritto fondamentale, sullo stesso piano della libertà, della vita, della salute; ogni altro valore costituzionale (tra cui l'esercizio dell'azione penale obbligatoria) non può,

si traduce in una sorta di obbligo mai verificato a condurre il sospetto alle sue estreme conseguenze, come se il sospetto

Il Senato voterà liberamente. Non è il mio linguaggio dire che non ci sto, però vorrei che voi vi domandaste che diritto avete di sottoporre un essere umano, certo nato a Casal di Principe, ma non per questo figlio di un Dio minore, a questo imbarbarimento. Il senatore Ciampi denunciava l'imbarbarimento della lotta politica in una bella intervista che ho letto,

per poi essere riconosciuto innocente tra dieci anni è come lasciarmi morire». Sono parole che bastano e avanzano per oppormi a che il diritto-dovere di indagare possa svolgersi senza limiti di tempo Concludo ricordando che nel 1993, in Senato, sul caso Andreotti mi trovai solo: non me ne vanto, né lo rimpiango. Mi premeva oggi, su un'altra vicenda di cosiddetto concorso esterno, esprimermi con analoga cultura delle garanzie e della libertà sottoponendovi queste considerazioni. Mi sembrava di doverlo a quest'Assemblea e a quel che essa significa per me. Se ci fossi riuscito, ne sarei onorato. Grazie!

Signore e signori del Senato, l'articolo 27 della Costituzione, secondo comma, recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Signore e signori del Senato, articolo 27, secondo comma, della Costituzione: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Articolo 27 della Costituzione, secondo comma, signore e signori del Senato: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». La Costituzione, all'articolo 27, secondo comma, recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». *(Applausi dal Gruppo PdL).* Il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione testualmente dice: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

il secondo comma dell'articolo 27 non è cambiato in questi attimi e recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

ha voluto citare un libro di Sciascia intitolato «Il contesto». Ebbene, proprio il contesto credo sia la guida per cui, pur avendo sottoscritto, io e la senatrice Poretti la mozione [1-00043, non parteciperemo al [Il contesto era quello dell'ottobre del 2008 in cui i radicali per la seconda volta occupavano la Commissione di vigilanza Rai perché si rispettasse la legalità costituzionale. Mi sarebbe piaciuto ascoltare in quei giorni un intervento, come quello poc'anzi offerto alla nostra Assemblea dal senatore Compagna, appassionato quanto sovrapponibile interamente ad uno Stato di diritto Il contesto odierno è fondamentalmente cambiato ed in parte evolve da ciò che era al centro di quella mozione che noi sottoscrivemmo, perché, all'interno del nostro movimento Radicali italiani, vi era chi riteneva opportuno chiedere che si ponesse la questione della qualità delle candidature ed anche delle nomine a Sottosegretario del Governo. Oggi siamo di fronte a una situazione in cui alla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati è stata richiesta la custodia cautelare in carcere per qualcuno che è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che - concordo pienamente con il senatore Compagna - non dovrebbe appartenere al diritto penale di *(Applausi dal Gruppo PdL).* Il problema è che i sospetti che erano al centro del contesto in cui sottoscrivemmo quella mozione oggi non si sono tramutati in prove e, quindi, risulta come minimo anacronistico chiedere oggi, a 13 mesi dal momento in cui si sottoscrisse quel documento

si potrebbe parlare a lungo degli aspetti giudiziari del caso Cosentino. Della tempistica di un'inchiesta fondata su accuse che risalgono ai primi anni '90, che diventa fascicolo giudiziario nel 2001, è pubblicizzata da «L'espresso» nell'autunno del 2008, con un'iscrizione nel registro degli indagati formalizzata il 12 febbraio 2009, una richiesta d'arresto cautelare firmata dal Pm dopo appena cinque giorni, e sottoscritta dal Gip dopo nove mesi, il tempo di una gravidanza. Si potrebbe parlare a lungo di un'indagine incubata in un enorme lasso di tempo, sistematicamente anticipata a mezzo stampa, sorprendentemente scadenzata in coincidenza con appuntamenti importanti della vita politica, e senza che mai Nicola Cosentino abbia avuto la possibilità di essere ascoltato. E ci si potrebbe chiedere, non senza fondamento, quali consapevolezze avessero indotto i colleghi dell'opposizione a sollecitare con un atto parlamentare le dimissioni del Sottosegretario al tesoro già nell'ottobre del 2008, quando Cosentino non era ancora formalmente indagato, e a dar conto delle accuse nei suoi confronti, per noi comuni mortali che non possediamo né scienze né conoscenze particolari, era stato solo qualche articolo del giornale «L'espresso». Si potrebbe parlare a lungo di un'ordinanza che Roberto Saviano ha definito «un trattato di antropologia e sociologia e non solo un documento giudiziario», e che, dopo averla compulsata, io definirei più un trattato di antropologia e sociologia che non un documento giudiziario. Di tutto ciò si potrebbe parlare a lungo, ma non è questa la sede per farlo. Oggi la maggioranza intende piuttosto affermare una cosa semplice: che non si piegherà al tentativo di trasformare l'Italia nella Repubblica dei pentiti. Ci siamo battuti perché non fosse l'iniziativa di qualche magistrato politicizzato a sovvertire la volontà del popolo sovrano, perché convinti che solo con un rapporto equilibrato fra giustizia e politica la politica può preservare la propria ragion d'essere e la giustizia la propria autonomia. A maggior ragione impediremo che a stabilire chi abbia titolo e chi no a far parte del Governo del nostro Paese siano le parole di un pentito, magari pure cocainomane o psichicamente infermo. noi rialziamo la bandiera del garantismo, che non è mai stata la bandiera dell'impunità. Collega Carofiglio, noi ci ricordiamo di Leonardo Sciascia e dei professionisti dell'antimafia. E ci soffermiamo a considerare quale grave precedente si vorrebbe stabilire attraverso il caso Cosentino da parte dell'opposizione, ivi compresa - e ce ne dispiace quell'UDC che pure sulla pelle dei propri esponenti ha giustamente tenuto duro sul principio inviolabile della presunzione di innocenza. *(Applausi lasciamo a Robespierre e ai suoi seguaci dei nostri giorni gli ideali astratti e assoluti di giustizia. Noi ci caliamo nel presente vivo, consideriamo il momento storico che stiamo vivendo. E abbiamo il coraggio di affermare che accedere oggi alla richiesta dell'opposizione, accettare che un'indagine basata sulle parole non riscontrate di qualche pentito debba comportare le dimissioni di un membro del Governo, inferirebbe un'ulteriore ferita al primato della politica e alla democrazia fondata sulla sovranità del popolo. E provocherebbe anche - voglio sottolinearlo - lo svilimento del ruolo dei collaboratori di giustizia, che da strumento investigativo nelle mani dell'autorità giudiziaria rischierebbero così di trasformarsi nei terminali di possibili ricatti politici, tanto più micidiali quanto più da parte del Parlamento si attribuisca a simili operazioni la garanzia di successo. Non ci nascondiamo dietro un dito, colleghi senatori. Oggi stiamo vivendo le prove generali per l'entrata in scena di Gaspare Spatuzza, che l'intensificarsi del rullo dei tamburi e l'iperattivismo dei corifei annidati in alcune Procure e in alcune redazioni di giornali preannunziano come imminente. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Se consentiamo che sia Gaetano Vassallo a decidere che Nicola Cosentino non possa sedere tra i banchi del Governo, cosa diremo al nostro popolo, al popolo italiano, quando altri pentiti, da altri palazzi di giustizia, cercheranno di riscrivere la storia del nostro partito, la storia del nostro leader, la storia del nostro Paese? Respingeremo stasera queste mozioni convintamente, e lo faremo anche per non rinunziare ad una speranza: quella di lasciare ai nostri figli un Paese finalmente normale.

Credo che con questo spirito, che è uno spirito laico e istituzionale, il Governo non possa non rassegnare un parere contrario ad entrambe le mozioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda che stiamo affrontando contiene in sé caratteri di estrema delicatezza perché richiama temi già svolti, che hanno impegnato la politica e la riflessione dell'opinione pubblica degli ultimi 20 anni e che interrogano il rapporto tra magistratura e classe politica e anche i fondamenti dello Stato di diritto. Io ho anche osservato, perché è doveroso farlo, i contenuti più immediati di questa vicenda, la sua specificità e alcune anomalie, che il collega Quagliariello ha rappresentato velocemente, anche rispetto alla tempistica di questa vicenda processuale. Questo accresce in noi, nel Movimento per le Autonomie, la forza delle ragioni che fanno prevalere l'esigenza di garanzia rispetto a qualsiasi altra esigenza. Inoltre, al di là del richiamo formale e solenne del senatore Longo ai principi costituzionali della presunzione di innocenza, siamo davvero convinti che l'iniziativa di una parte processuale, qual è il pubblico ministero, debba essere rispettata e osservata con grande attenzione, ma che essa non costituisca la definizione piena di una procedura giurisdizionale. Vi è una fase che prevede e pretende riscontri; vi è una fase

serio le garanzie che il nostro sistema giurisdizionale appresta per qualsiasi cittadino. Per queste ragioni, noi riteniamo che le mozioni di revoca presentate nei confronti del sottosegretario Cosentino debbano essere respinte da questo

che alcuno debba interpretare questo atto come un privilegio di casta e come una forma di copertura per le responsabilità e senza costituire alcuna forma anticipata di immunità, il Senato deve difendere i principi di garanzia

e di garanzia che il nostro ordinamento deve apprestare a tutti i cittadini, e anche agli esponenti dell'Esecutivo, mi consentirete - siccome non amo sfuggire anche a una riflessione di merito politico

l'esigenza di trasparenza e di rigore, oltre che l'assenza di qualsiasi sospetto, rappresentano condizioni essenziali per garantire il prestigio delle istituzioni su un'area importante qual è il Mezzogiorno del Paese, dove la sfida alla criminalità costituisce impegno primario del Governo. Per questa ragione, con grande serenità,

Signor Presidente, onorevoli senatori, insieme ai colleghi del Partito Democratico il 22 ottobre del 2008 abbiamo predisposto e sottoscritto una mozione che viene oggi discussa in un testo identico a quello di un anno fa. È questa la ragione per la quale, lo anticipo, voteremo contro la mozione presentata dai colleghi dell'Italia dei Valori, e di una concezione diverse del rapporto che deve esserci tra politica e magistratura. Abbiamo sentito questa sera in quest'Aula tante importanti opinioni - alcune anche parecchio condivisibili -

non c'è alcuna somiglianza, né sul piano politico, né su quello istituzionale, né sul piano della statura delle persone, lo dico con il dovuto rispetto. Credo che quando si arriva a tanto

quando il Parlamento, ancorché con i limiti di cui forse qualche giorno parleremo, si pronuncia su queste vicende, lo fa nell'esercizio di una prerogativa e di una funzione costituzionalmente rilevante, che non può essere derubricata a privilegio di casta.

un ruolo, che è quello del Senato, che è chiamato qui a discutere di una mozione che ha un rilievo di natura squisitamente politica e che da un anno segnala una questione di opportunità legata alla funzione specifica di Governo che l'onorevole Cosentino disimpegna e non ad un giudizio anticipatorio, né sul piano giudiziario, né meno che mai sul piano morale, delle qualità umane e politiche del deputato Cosentino. Ma credo sarebbe stato anche più opportuno affrontare questa riflessione evitando di far seguito ad una decisione dell'autorità

Ma noi non stiamo discutendo di questo. Noi stiamo discutendo del fatto che è necessario, in questo Paese e in questo Parlamento, un sistema di regole minime e condivise, che disciplinino il rapporto e che consentano a chi disimpegna determinate funzioni di farlo con serenità, senza mettere in imbarazzo l'istituzione che rappresenta o il partito e il Gruppo parlamentare che rappresenta. Un minimo di regole condivise, che prescindano dalla vicenda giudiziaria, le dovremmo trovare. Altrimenti, come spesso è avvenuto ed avviene nel nostro Paese in questa logica pseudobipolarista, si condanna o si assolve a seconda del luogo politico in cui l'interlocutore si trova.

anche in terre molto particolari, come la Sicilia. Io credo che buona norma avrebbe voluto che questa maggioranza avesse preso in considerazione questa mozione un anno fa, segnalando all'onorevole Cosentino l'opportunità di fare un passo indietro dall'esercizio delle sue funzioni, in attesa che queste vicende venissero chiarite. Non era invece il caso di accedere alla tesi di anteporre a questo minimo codice codice deontologico una serie enorme, ingiustificata ed inappropriata di considerazioni sofisticate, intelligenti ed acculturate (non so cosa altro dire per riempire di complimenti chi le ha fatte), ma che tuttavia non hanno nulla a che vedere con il caso di cui ci stiamo occupando. Quello di cui ci stiamo occupando è il caso di un personaggio che, fino a prova del contrario e fino a definizione degli eventuali giudizi, si presume essere innocente (così come dice la Costituzione), ma che al contempo si trova a svolgere una funzione delicata, essendo responsabile presso il Ministero dell'economia di flussi consistenti di finanziamento, che riguardano

di suggerire una valutazione di opportunità in merito all'assoluta incompatibilità, sul piano politico, dello svolgimento di quell'incarico con le vicende che riguardano l'onorevole Cosentino (che ci auguriamo venga fuori presto

vorrei dire, concludendo, al senatore Quagliariello, io credo che non sia opportuno

Credo che recuperare quel senso delle istituzioni e quella tradizione farebbe bene a tutti, soprattutto a quelli che utilizzano questo sistema a giorni alterni. Chi vi parla lo sa, perché vive in una terra in cui questa doppia verità è stata usata a mani piene e a mani basse,

Presidente, colleghi, signori del Governo, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato, fin dall'ottobre 2008, una mozione per avviare con immediatezza le procedure di revoca dell'onorevole Nicola Cosentino da sottosegretario di Stato. Ricordo al senatore Compagna, leggendo il decreto di nomina pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2008, n. 178, che il Sottosegretario di Stato ha competenze sul dipartimento del tesoro, sulle questioni relative alle provvidenze in favore delle imprese radiofoniche e televisive e sulle questioni concernenti le sedute del CIPE.

per difendersi in modo libero dai fatti che gli venivano contestati. Egli avrebbe così, da cittadino, ancorché non più da componente dell'Esecutivo, dato maggior credibilità alle istituzioni, evitando un corto circuito e un inutile arroccamento su privilegi e guarentigie di cui i cittadini hanno le tasche piene.

intorno non fosse avvenuto. Il 9 novembre 2009, però, la «pratica Cosentino» si arricchisce della richiesta di custodia cautelare in carcere, non per una bazzeccola ma per una contestata violazione degli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale, ovvero concorso esterno in associazione di stampo camorristico. Non intendiamo entrare nel merito della vicenda giudiziaria - che è demandata alla magistratura - e nemmeno nella competenza dell'altro ramo del Parlamento secondo la procedure previste dall'articolo 18 del Regolamento della Camera, procedure che peraltro non si sono ancora concluse. Neppure noi

sul tappeto, all'attenzione dell'Aula e della pubblica opinione, il problema del rapporto tra istituzioni e cittadini che coinvolge il prestigio e la dignità di tutto il sistema Italia. Sappiamo tutti del rapporto sempre più difficile tra il Paese reale e il mondo della politica e delle istituzioni, una spaccatura che va ampliandosi proprio per la protervia con cui i potenti, sempre più spesso prepotenti, cercano di tutelare se stessi e i loro amici a dispetto di qualsiasi e più elementare senso civico. Assistiamo a leggi *ad personam*, alla tutela dei bancarottieri e dei banchieri che hanno turlupinato e spesso truffato i risparmiatori per arrivare, infine, al cosiddetto ammazza-processi, già in arrivo in quest'Aula, per dare il salvacondotto definitivo e a vita al presidente del Consiglio Berlusconi, alla faccia dell'articolo 3 della Costituzione e alla faccia di quello che viene ormai indicato come il provvedimento che assesterà un colpo definitivo alla giustizia italiana. Ebbene, nonostante questa conclamata e del tutto giustificata avversione dei cittadini nei confronti della classe politica, anziché presentare le proprie dimissioni e nonostante lo scudo protettivo che ha come parlamentare, l'onorevole Cosentino continua ad occupare imperterrito la sua postazione.

Ragioni di opportunità e perché no, di ragionevole precauzione avrebbero dovuto indurre il Governo ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini per così gravi motivi, espressivi di una collusione tra politica e sodalizi criminosi - certamente non stiamo dando un giudizio prognostico - potesse continuare ad esercitare la propria funzione di governo, peraltro in un ruolo assai delicato che riguarda , tra l'altro, la funzionalità dello dello stesso Esecutivo. Dato che queste dimissioni spontanee che gli abbiamo richiesto in base al senso di responsabilità non sono arrivate, probabilmente vale la pena ricordare cosa succede e cosa è successo nei Paesi dell'Europa, e non solo. Nel 2005 il Ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria francese si dimise perché aveva avuto in fitto gratis un appartamento di 600 metri quadri e disse: «riconosco di aver commesso errori di giudizio». Nessun reato!

Il 24 gennaio 2008 in Gran Bretagna rassegna le dimissioni il Ministro del lavoro, in seguito alla mancata dichiarazione di donazioni ricevute per la campagna elettorale. Nel 2008 in Perù il Presidente accetta le dimissioni del Premierin seguito ad uno scandalo sulle intercettazioni telefoniche, il cui processo non si è ancora concluso. Nel 2008 il portavoce del Governo greco si dimette per uno scandalo che non lo coinvolge direttamente. Anche se egli nega qualsiasi addebito, lascia l'incarico per non pesare sull'attività di Governo. Infine, il 18 maggio 2009 lo *Speaker* della Camera dei Comuni inglese si è dimesso in seguito allo scandalo dei rimborsi spese ai parlamentari. Anche se di quegli imbrogli Martin non si è mai personalmente macchiato, se ne giudica egli stesso responsabile e ritiene di rassegnare le dimissioni. Qui nessuno vuole inseguire giustizialismi di sorta; nessuno vuole negare la garanzia che hanno tutti i cittadini e nemmeno la si intende negare al sottosegretario Cosentino. Ma egli bene farebbe dinanzi al Paese, assumendosi la responsabilità di difendersi - come egli sono sicuro farà - a dimettersi, dando davvero credibilità, dignità e maggior prestigio al

le due mozioni presentate dall'Italia dei Valori e dal Partito Democratico, seppur diverse nei toni e nelle premesse, convergono verso un unico obiettivo sostanziale: la sfiducia individuale nei confronti di un sottosegretario, l'onorevole Cosentino. Non entreremo nel merito del procedimento penale condotto dalla procura della Repubblica di Napoli. Facciamo solo rilevare che questo procedimento pende, per la fase di indagini preliminari, dal 2001 2001 e che trae origine da deposizioni di testimoni pentiti ascoltati nel 1994. Dico che questo ci fa riflettere - vedo il sottosegretario Caliendo sul discorso del processo breve e sulla durata ragionevole dei processi. Per fortuna, abbiamo escluso le indagini preliminari dal disegno di legge, altrimenti l'accusa sarebbe stata quella di aver voluto coprire il caso Cosentino anche con il disegno di legge sul processo breve. Né abbiamo intenzione di interferire con i lavori della Giunta della Camera di deputati, che proprio oggi ha rigettato la domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'onorevole Cosentino. Anche qui un dibattito articolato: sarà l'Assemblea della Camera a decidere definitivamente. Non è neanche nostra intenzione analizzare la figura giuridica del Sottosegretario, ma anche su questo aspetto inviterei i colleghi di sinistra a rileggere un saggio di Leopoldo Elia del 1967, che chiarì perfettamente qual è la funzione vicaria di un Sottosegretario, che non esercita funzioni di governo, se non nei limiti della delega che gli conferisce il Ministro. La legge del 1988 ha confermato questa impostazione, affermando che i Sottosegretari coadiuvano il Ministro, che giustamente la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico spettano esclusivamente al Ministro. D'altronde si tratta di un principio contenuto anche nella Costituzione. esame sono un'iniziativa del tutto irrituale dal punto di vista istituzionale e parlamentare; è un inutile - e direi anche goffo - tentativo di anticipare una campagna elettorale per le elezioni regionali che si svolgerà tra pochi mesi e che vedrà, nell'ambito degli argomenti di critica politica, sicuramente anche questi aspetti, che però non dovevano trovare spazio in una mozione in Parlamento. Contestiamo quindi l'ammissibilità di queste due mozioni di sfiducia, due mozioni di sfiducia, che partono da presupposti del tutto sbagliati dal punto di vista parlamentare e istituzionale. Fare, come fa la mozione dell'Italia dei Valori, un salto logico con l'affermazione secondo cui - riporto testualmente - «il rapporto fiduciario tra Camera e Governo deve considerarsi direttamente trasposto anche in riferimento ai Sottosegretari di Stato», significa dimenticare volutamente le regole della Costituzione, gli articoli 92, 94 e 95, o meglio piegare queste regole a puri scopi propagandistici, con buona pace di tutti i richiami che in quest'Aula vengono spesso fatti a sproposito alla nostra Carta fondamentale. La mozione di sfiducia individuale nei confronti di un Sottosegretario, indipendentemente da ogni altra considerazione in termini di opportunità e di merito, appare quindi assurda alla luce della Costituzione e della prassi parlamentare di 50 anni di storia repubblicana. Non esiste una responsabilità politica individuale di un Sottosegretario, ma esiste una responsabilità politica del Governo e del Ministro. La sfiducia individuale del Sottosegretario, se approvassimo queste mozioni, comporterebbe il riconoscimento al Sottosegretario di un potere di indirizzo politico autonomo, incostituzionale: un vero e proprio strappo alla Costituzione. Quale parametro poi potremmo utilizzare per esprimere un giudizio di responsabilità politica che porta alla rimozione di una persona dalla carica di Sottosegretario? Il Sottosegretario non ha un suo programma di governo, non espone in Parlamento le sue linee programmatiche; rimarrebbe quindi solo un parametro legato alle qualità e ai comportamenti personali. Qui il piano, colleghi, diventa davvero scivoloso; se venisse accolta questa impostazione, allora dovremmo passare al setaccio la vita individuale e i comportamenti di tutti i componenti del Governo e il giudizio di responsabilità diventerebbe un giudizio etico e morale. Ma forse, poi, alla fine, è davvero questo l'intendimento delle due mozioni. sentito dal collega Carofiglio l'equazione indagato-indegno-dimissioni: questa è la teorizzazione del governo dei giudici, espressa in maniera molto chiara, che noi rifiutiamo. I Sottosegretari operano in virtù di una delega specifica, e le responsabilità di questa delega competono al Ministro, unico componente di organo politico sorretto dalla fiducia politica del Parlamento; i Sottosegretari non hanno alcun rapporto fiduciario con queste Camere. Questa iniziativa parlamentare, al di fuori del sistema costituzionale, non può trovare in alcun modo il nostro consenso; per questi motivi esprimeremo un voto contrario.

È un profilo che riguarda non tanto l'aspetto costituzionale, su cui si è soffermato appena adesso il collega della Lega, quanto la coerenza logica. Mi spiego molto brevemente.

dovrà essere corredata da riscontri individualizzanti», in mancanza dei quali le dichiarazioni rese non possono essere considerate dimostranti la colpevolezza. Sono d'accordo con questo punto, che è altamente tecnico, e non è un caso che tale mozione sia firmata da illustri senatori magistrati: Finocchiaro, D'Ambrosio, Della Monica, Casson, Maritati ed altri che non conosco (c'è anche il senatore Latorre

torno a richiamare questo elemento tecnico ed a rivolgermi proprio a questi magistrati, colleghi per i quali ho grande stima anche per aver avuto con loro confessabili, ancor prima che fossero magistrati. Vorrei ricordare a loro ed ai colleghi che mi ascoltano che qualche legislatura fa

Quella battaglia non ebbe alcun esito, l'articolo 192 non fu modificato e la maggioranza di sinistra non volle cambiarlo. La conseguenza è che abbiamo avuto procedimenti giudiziari di tipo solipsistico, dove la dichiarazione di un pentito viene riscontrata con la dichiarazione di un secondo pentito, quella del secondo con il terzo, fintantoché l'ultimo pentito dichiara esattamente quanto ha dichiarato il primo della catena ed il cerchio si chiude. La conseguenza è che ci sono state condanne importanti, anche con apparente valore storico, ottenute sulla base di dichiarazioni di pentiti, che poi sono state messe in discussione sulla base di dichiarazioni di altri pentiti.

che si impegna il Governo ad invitare il Sottosegretario a rassegnare le dimissioni, non si debba premettere che il Senato impegna il Governo

Senatore Pera, questa Presidenza ha ritenuto ammissibili tali mozioni che, seppur al proprio interno possono mantenere profili di presunta contradditorietà, attengono alla stesura ed all'impostazione di coloro i quali le hanno redatte. Per quanto ci riguarda, si tratta di rapporto interorganico: sono mozioni con cui si chiede al Senato di invitare il Governo ad assumere determinate scelte in ordine ad alcune nomine di Governo.

anche il presidente Pera ha ritenuto di prendere la parola per rilevare l'inammissibilità di una mozione - non di un ordine del giorno, mi dispiace doverlo correggere - che la Presidenza del Senato aveva evidentemente ritenuto ammissibile, visto che ormai la stiamo discutendo

nel dettaglio sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che richiamano i suoi rapporti penalmente rilevanti con il *clan* camorristico dei casalesi. Mi limito a ricordare che si tratta di una delle associazioni criminali più pericolose e sanguinose della nostra Repubblica.

per me sacrosanto, ma che non sempre vedo osservato dalla maggioranza - di rispettare con il massimo scrupolo la divisione dei poteri

Anche per questo motivo, i 24 senatori che hanno firmato la mozione su cui sto chiedendo il voto favorevole del Senato

non abbiamo integrato il testo con il seguito che la vicenda ha avuto, vicenda ha avuto, perché la questione di cui dobbiamo discutere oggi riguarda esclusivamente l'opportunità che un parlamentare inquisito per rapporti con la camorra,

a quanto di competenza della Camera dei deputati. Noi ci occupiamo di altro. Oggi i senatori con il loro voto possono far capire al Paese di avere coscienza dei limiti e della misura del loro potere e dimostrare qual è oggi il nostro senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni. Oggi il Senato con il suo voto può restituire dignità al Parlamento. Parlamento. Chi come noi ha l'onore di sedere in Senato non può non sentire quotidianamente il peso del giudizio negativo dell'opinione pubblica sui privilegi veri o presunti come ha ricordato stamattina il presidente Gasparri - della politica e degli eccessi dei comportamenti di tanti uomini politici. Noi non possiamo ascoltare le proteste della gente, sentirne il malumore e far finta di nulla; non possiamo rimuovere né considerare le nostre responsabilità nella pericolosa, ma purtroppo comprensibile, diffusione di sentimenti di antipolitica e di sfiducia nelle istituzioni.

il deputato Fabio Granata, in un'intervista molto amara ma profonda, ha detto che chi crede nella legalità, nell'antimafia e nella giustizia, chi ha senso dello Stato viene guardato come un appestato. Non lo dico io, ma un deputato del centrodestra.*(Commenti Sono giudizi che faremmo molto male a sottovalutare, perché nella società italiana c'è un visibile, chiarissimo, palpabile precipitare di tenuta morale, c'è un diffuso rifiuto di ogni senso del limite, c'è una ostentata volgarità nell'uso del potere che sta danneggiando la nostra credibilità e riducendo il nostro Paese a zimbello della comunità internazionale. Oggi noi possiamo fermare questa deriva, ma lo possiamo fare solo se riusciamo a dare una risposta alla domanda di rispetto delle istituzioni e dello Stato che ci rivolgono i cittadini onesti. Il Senato deve riconoscere all'onorevole Cosentino, come a tutti i cittadini, il diritto di essere considerato non colpevole fino alla condanna definitiva; ce lo ha ricordato prima il senatore Longo al quale voglio solo dire che non sto

a favore della mozione che stiamo discutendo, il Senato deve affermare il fondamentale principio di etica politica che vieta a un cittadino nei cui confronti la magistratura ha emesso un ordine di custodia cautelare

concordo con lui, ma solo se questo argomento non viene usato per screditare il lavoro difficile e rischioso della magistratura. Noi non stiamo parlando di pentiti, senatore Quagliariello, ma di decisioni legittime dell'autorità giudiziaria,

che il suo partito deve votare contro le mozioni con voto preventivo, come forma di cautela rispetto a future analoghe iniziative nei confronti del presidente Berlusconi. Lei lo ha detto esplicitamente e io le rispondo

quando comunque riguardano le persone. Quel "comunque" fa la differenza tra noi e la Camera dei deputati. Il nostro Regolamento è chiaro: tutte le votazioni che comunque riguardino persone possono avere il voto segreto. Oggi, però, noi non chiediamo il voto segreto

ed anche la comunità internazionale (che da tempo sta seguendo l'etica della nostra politica) possano conoscere il nome ed il cognome dei parlamentari che difendono l'onore, la dignità ed il decoro del Governo italiano. Per tale motivo, io chiedo un voto palese. *(Applausi dai Gruppi PD e

i senatori del Popolo della Libertà non hanno avuto difficoltà, anzi per certi versi hanno voluto che questo dibattito si svolgesse. Lo hanno voluto fortemente qui, nell'Aula del Senato, perché la stagione dei pentiti dal credito preventivo che ad essi si vuol dare ci preoccupa. La nostra preoccupazione vale quanto la faciloneria di alcune procure ad accreditarli come oracoli, al punto tale che il senatore Zanda parla di rinvii a giudizio che ancora non ci sono stati. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Questo è il modo con cui intendete la giustizia! Questa è la verità dei fatti! Se vi fosse stato bisogno di dimostrare quanto siano mendaci alcuni argomenti, il senatore Zanda, forse per imperizia, ce ne ha offerto un altro: non vi è alcun rinvio a giudizio. Spatuzza contro Dell'Utri, Vassallo (già descritto giustamente dalle cronache come cocainomane e persona dalla dubbia sanità di mente) contro Cosentino, e vi sono tanti altri pentiti pronti a formulare accuse contro chiunque; si accreditano come fonti di ogni azione penale. Falcone perché noi siamo dalla parte della magistratura, ma sappiamo scegliere i modelli a cui ispirare il nostro rispetto verso la magistratura, e Falcone, Borsellino e molti altri sono memorie carissime di tutta la Repubblica italiana e certamente nostre! per Falcone non doveva essere così: ogni dichiarazione dei collaboratori e dei pentiti andava sottoposta a verifiche e controlli e poi ad ulteriori verifiche e controlli, senza mai consentire agli elementi di fatto indicati in tali dichiarazioni di contraddire attente e documentate compatibilità di luogo, di tempo e di azione. Poi Falcone fu ucciso, fu sterminato in quell'orrenda strage. Ricordo gli argomenti ed i sentimenti con i quali era stato avversato in seno alla magistratura, perché ancora oggi girano in Parlamento coloro che hanno accusato Falcone di ogni nefandezza: ricordiamo benissimo

oggi nella magistratura organizzata e - ahimè! - a volte anche nello stesso Consiglio superiore della magistratura finiscono per prevalere altri criteri di azione e di valutazione; ma l'insegnamento su come utilizzare o non utilizzare i pentiti per noi resta valido anche se qualcuno lo ha fatto cadere in desuetudine. È arrivata poi la stagione del "casellismo" e ve ne è stato un uso come «arma impropria». Nel corso della XIV legislatura è stato presentato dal senatore Iannuzzi e da 100 senatori un disegno di legge che proponeva una Commissione parlamentare d'inchiesta sul pentitismo e sui riflessi

Oggi mi torna in mente la vicenda degli anni Novanta quando l'allora procuratore di Palermo, di fronte al caso Di Maggio, parlò della gestione dinamica dei pentiti. Io ricordo bene quella vicenda: c'era un pentito, Di Maggio, cioè un esponente della mafia che si considerò pentito e venne rimandato a casa, in Sicilia. Maggio, essendo libero? Sterminò i capi delle cosche rivali, approfittando di questa generosità. Era pentito, ma non abbastanza da privarsi del gusto di qualche regolamento di conti.

sono gli inconvenienti o i frutti della gestione dinamica dei pentiti. Ossia: noi lo consideriamo pentito, lo mandiamo a casa e ammazza un po' di gente; invece di andare in palestra o di fare *footing*, si scaricava secondo le consuetudini delle sue cosche e del suo stile. Su questa vicenda vorremmo che qualcuno rispondesse!

criteri di opportunità. Devo dire che abbiamo ascoltato con sorpresa anche l'intervento del senatore D'Alia, dal quale ci saremmo attesi maggiore equilibrio, attenzione e cautela, anche alla luce

Poi mi chiedo, caro senatore Zanda, se le indagini risalivano al 1990, a decenni prima, come mai le decisioni arrivano alla vigilia delle elezioni regionali che si preannunciano una catastrofe per la sinistra campana della spazzatura, degli scandali e delle tante inchieste?! *(Applausi dopo! Se dimissioni e arresti erano necessari, forse servivano vent'anni fa. In vent'anni, se uno fosse stato un criminale, quanti reati poteva compiere? Invece adesso ci sono le elezioni e quindi c'è questa solerzia.

Potremmo chiedervi: chi gestiva a Castellammare di Stabia il tesseramento del Partito Democratico, dove vi siete trovati iscritte persone che sparavano *(Applausi dal Gruppo* *PdL)* e persone che sono state uccise perché forse qualcosa non funzionava?

Vorrei ringraziare il ministro Maroni, i sottosegretari Mantovano e Nitto Palma e tutti coloro che sono al Viminale perché il «modello Caserta» lo si deve a questo Governo, che ha spazzato via intere cosche in tutte le parti d'Italia e soprattutto in Campania e nella provincia di Caserta *(Applausi dai a vantaggio ed onore del nostro Governo e della nostra maggioranza! E allora, continueremo anche nella riforma della giustizia. Abbiamo varato quella del processo civile e abbiamo approvato tante leggi. Stiamo discutendo di processo penale e di una giustizia con tempi più rapidi, ma non per tutti: per camorristi e mafiosi le nostre proposte, a differenza delle vostre, non pongono limiti di tempo all'azione della magistratura! Ecco, cari colleghi, i modelli: c'è chi sceglie Spatuzza e Abu Omar; noi scegliamo i valori della legalità repubblicana. Ed è per questo che voteremo no alle vostre mozioni.

resti agli atti. Non parteciperò al voto per sottrarmi a questo clima che stiamo vivendo e per tre ragioni particolari. La prima è che questa mozione era più giustificata nell'ottobre 2008 quando fu presentata: non vi era un procedimento giudiziario in corso, o almeno non se ne aveva notizia. Oggi vi è una procedura in corso: la Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione all'arresto e penso che questa mozione avrebbe dovuto essere ritirata. Il secondo punto è che non mi sento in coscienza di esprimere un giudizio, perché questo sarebbe - al di là della lettera della mozione e della volontà dei proponenti - di colpevolezza. Sento oggi di dire questo, anche per poter condurre in modo più limpido la battaglia contro quella che considero una manomissione della giustizia e del diritto, che maggioranza e Governo stanno cercando di mettere in atto. Il terzo punto, infine, è che non intendo alzare la palla ai senatori Gasparri e Quagliariello, che dipingono una notte della giustizia nera in cui tutte le vacche sono indistinte, una notte in cui non ci sono verità da conoscere e da verificare, ma un complotto, anzi una serie ininterrotta di complotti, passati, presenti e soprattutto futuri, da denunciare e da mettere a tacere.

Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

limite temporale il momento fino al quale si permane in attività lavorativa. Va da sé che, per una donna che spesso entra ed esce dal lavoro, ripetutamente nel corso della vita, si pone il problema della ricostruzione della propria carriera lavorativa e del recupero dei contributi figurativi per il periodo di congedo, alla vigilia del pensionamento. L'introduzione di questo limite temporale è l'ennesimo segno di discriminazione nei confronti delle donne e delle penalizzazioni a cui esse sono sottoposte in relazione alla loro funzione riproduttiva.

Il punto maggiormente critico riguarda la definizione degli aventi diritto (coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado). Riteniamo che la platea degli aventi diritto sia troppo ristretta

Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato hanno obbligato l'INPS a rivedere e adeguare i criteri adottati in merito all'accertamento dei requisiti. Non di «continuità» e di «esclusività» dell'assistenza offerta dal lavoratore alla persona con disabilità grave si deve parlare, ma di «sistematicità e adeguatezza». Se lo scopo della legge è quello di non privare mai il disabile di affetto e assistenza, ove il genitore congiunto o parente avente diritto possa trovarsi in condizione di non poter provvedere da solo all'incombenza, una interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un'altra persona possa sostituire momentaneamente almeno l'avente diritto originario. Per questo chiediamo di sopprimere l'articolo 18.

potuto cogliere l'opportunità di introdurre una disciplina più coerente con la situazione reale delle famiglie. Talvolta la nascita di un figlio

18.5 proponeva l'eliminazione del limite di un solo genitore per i permessi di assistenza a persone affette da handicap grave.

verso questi emendamenti: di ciò li ringrazio perché gli fa onore. L'emendamento 18.9 è stato poi cancellato nonostante mirasse a rendere semplicemente più elastica ed efficace la fruizione dei tre giorni di permesso al fine di garantire una assistenza ponderata sugli effettivi disagi di un figlio disabile. Questi emendamenti oggi sono ripresentati in Aula.

senatore Divina.

in tema di certificazione della disabilità, le informazioni cui fa riferimento il senatore Divina sono già disponibili: le commissioni di valutazione rendono evidenti le condizioni di grave

che, per coerenza, anche il 18.10, che dispone esattamente la stessa norma su un altro punto dell'articolo, richiederebbe analoga valutazione.

le norme sui provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni introdotte nel testo unico del cosiddetto decreto Brunetta. A parte le considerazioni sul merito delle norme introdotte dal decreto Brunetta, da cui emerge chiaramente la volontà punitiva del legislatore nei confronti del lavoratore, l'imposizione di tali norme e del rigido meccanismo in esse contenuto all'intero settore privato, senza alcuna distinzione, appare secondo noi arbitrario e irragionevole. Pertanto, invito il relatore ed il Governo ad accogliere la nostra richiesta di sopprimere l'articolo 19. Presidente, chiederei per un momento l'attenzione del relatore. L'emendamento 19.201 è stato presentato per rendere evidente che

Ghedini, tant'è vero che ho presentato l'emendamento 19.400. In realtà, il riferimento alla norma preesistente riguardava cinque

reca disposizioni concernenti il controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali relative alla disciplina legislativa in materia di lavoro, di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

non solo i diritti dei lavoratori e delle imprese, ma addirittura la capacità e il potere di controllo del giudice sul caso. Infatti, il comma 1 - su cui poi si interviene proponendone la soppressione con stabilisce che «il controllo giudiziale», laddove vi siano le clausole generali, «è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità». Questo contrasta con il criterio secondo il quale il giudice ha sempre l'obbligo di accertare la conformità o no del fatto alle norme di legge: non è solo un controllo di pura legittimità. E non può esimersi,

al comma 2, esso prevede addirittura che nella qualificazione giuridica del contratto il giudice venga vincolato non alla legge, ma alla valutazione delle parti, le quali, magari, anche in sede di certificazioni si sono accordate. È una cosa veramente strana perché si tratta della lesione di un principio generale: il giudice non può subire vincoli e condizionamenti dall'accordo delle parti nella qualificazione del contratto. Il giudice deve gli derivano unicamente dalla legge. Tutte le parti hanno il diritto di andare dal giudice a far valere i loro diritti,

il comma 3 vorrebbe costringere il potere di valutazione soltanto alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di maggior rilievo. Questa è una cosa ancora più strana, perché tale formula lede i principi fondamentali dell'interpretazione delle norme. Se le norme devono avere un carattere vincolante, e quindi non consentono al giudice di interpretare la legge, le tipizzazioni cui si fa riferimento sono contro il dettato costituzionale; al contrario, se invece si intende soltanto ammettere che il giudice può utilizzare queste tipizzazioni come elementi illustrativi della realtà, la norma è del tutto inutile, perché questo già succede, già lo fanno i giudici e già lo dice la Corte di cassazione. Per questo motivo con l'emendamento 23.8 si propone in via subordinata di sopprimere

chiederei ai colleghi un po'di attenzione, perché l'articolo di cui stiamo discutendo attiene ad una materia caldissima e delicatissima: quella del controllo giudiziale sui licenziamenti.

quindi un errore di metodo specifico nell'affrontare la materia in questo modo frammentario e oltretutto e oltretutto in un contesto confuso come quello di questa legge. Andando però al merito di questa norma, vorrei avvertire i colleghi che

ancora più incisivo e limitativo della libertà d'impresa di quanto non sia l'assetto della disciplina attuale. Il terzo attuale. Il terzo comma di questo articolo prevede che nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che «delle fondamentali regole del vivere civile» (ma questo non ci sarebbe nessun bisogno di dirlo, perché ovviamente qualunque giudice della Repubblica deve sempre tener conto delle fondamentali regole del vivere civile), anche dell'"interesse oggettivo" dell'"interesse oggettivo" dell'impresa. Ciò non significa soltanto che il giudice può sindacare le scelte dell'imprenditore, ma addirittura che esiste un interesse oggettivo oggettivo dell'impresa diverso dall'interesse soggettivo dell'imprenditore e ad esso sovraordinato. Tale concetto era stato introdotto nel nostro ordinamento in epoca corporativa, ma è stato largamente e compiutamente superato dalla cultura giuslavoristica successiva. Capite che votando questa norma voi addirittura legittimate il giudice del lavoro a farsi interprete

sensatamente pensare di reintrodurre nel nostro sistema. Questo riapre un capitolo giurisprudenziale pericolosissimo per tutti: per il sindacato da una parte, ma prima ancora per la libertà d'impresa.

che il giudice debba attenersi alla volontà negoziale delle parti circa la qualificazione del rapporto equivale a dire che il giudice deve attenersi al *nomen iuris*, cioè all'etichetta che le parti hanno hanno voluto dare al rapporto. Se di questo si tratta, la norma è palesemente incostituzionale. La Corte costituzionale ha più volte ribadito

"salvo il caso di erronea qualificazione del contratto" delle parti stesse. Se, però, il giudice deve tenere conto della loro volontà salvo che quest'ultima sia erronea,

evitare di fare pasticci e di complicare la vita all'intero sistema di relazioni industriali con una norma malfatta che o è inutile, o va nella direzione opposta a quella per la quale si è voluto dettarla.

del diritto delle parti, cioè sia del datore di lavoro o titolare dell'azienda che del prestatore d'opera, lavoratore subordinato; si tratta di due valenze importanti da mettere a sistema e a cui far trovare un punto di equilibrio.

il problema non è superfluo da affrontare o da porre. In effetti, il giudice si trova a dover decidere se sussistano i presupposti di fatto non soggettivi nel valutare l'interesse dell'azienda o dell'organizzazione. Se ci si dovesse rimettere all'interesse soggettivamente valutato o percepito da parte del titolare dell'azienda o dell'organizzazione, si entrerebbe in una materia in cui la soggettività ha confini illimitati; infatti, io potrei ritenere che l'interesse dell'azienda o dell'organizzazione si estenda fino a certe scelte commerciali, organizzative di ritmi e tipizzazioni dei modi di resa della prestazione di lavoro, un altro imprenditore o dirigente dell'organizzazione potrebbe avere soggettivamente una visione completamente diversa. Nel momento in cui scatti la controversia (perché siamo in una materia di contenzioso), che cosa facciamo? Rimettiamo al giudice

ma perlomeno si offre un criterio di riferimento e un parametro al giudice, che ha dato - ahimè - infiniti esempi di soggettività quando non addirittura di arbitrio nella molteplice giurisprudenza cui abbiamo assistito. Questa parola Questa parola in qualche modo lo costringe a un criterio di riferimento che varchi la soggettività. Capisco che stiamo parlando di una distinzione in molti casi capillare,

Quando si osserva che ciò sarebbe in contraddizione con il caso di erronea qualificazione del contratto, in realtà si dichiara una cosa non esaustiva, non esauriente, non chiarificatrice, perché in effetti il giudice qualificherà il contratto a misura della volontà sostanziale delle parti. Se le parti hanno dato un *nomen iuris* aberrante a quello che, nella loro volontà, esprimono nelle modalità del rapporto come qualcosa che corrisponde a tutt'altro istituto, ad altro rapporto contrattuale

La verità è che si tratta di una materia che nessuna normazione riuscirà mai in maniera esaustiva a rendere tranquilla *a priori* rispetto a un'eventuale controversia che sorga. Si tratta tuttavia di due avvicinamenti all'obiettivo, che riterrei meritevoli di attenzione e di pregio.

questioni assai delicate e complesse, ma l'articolo 23 contiene una scelta ben determinata e ben precisa. Sappiamo che spesso si rimprovera al giudice una discrezionalità che spesso sconfina nell'arbitrio o una mancanza di tipizzazione di fattispecie che spesso consente ed obblighi a ricorrere ai principi generali che possono avere soluzioni tra le più svariate e variegate. Sicuramente molti di voi ricorderanno una sentenza degli anni Settanta del pretore di Milano, che stabilì che il dipendente che aveva un rapporto amoroso con la moglie del datore di lavoro non costituiva una causa di licenziamento, né un giustificato motivo, perché il rapporto si consumava al di fuori dell'orario di lavoro. Sono queste le conseguenze che possono determinarsi laddove non vi sia una normativa precisa, che tipizzi in maniera

la libertà di contrarre. È indubbio che i contratti di lavoro abbiano natura privatistica ed è indubbio che le parti, al di fuori di certi limiti che attengono all'ordine pubblico, al buon costume e alle norme imperative, abbiano la facoltà e il potere di fissare qualsiasi fattispecie e di allargare i confini del loro contratto. è dato spazio a quell'autonomia alla quale ho fatto riferimento. E non è un problema di *nomen iuris* tanto è vero che è data al giudice la possibilità di modificare il *nomen iuris* laddove, attraverso le parti, si giunga ad un'erronea qualificazione del rapporto. Allora è come disegnare confini ben precisi, indicando una scelta che serve a dare maggiore certezza anche in ordine alle politiche industriali,

di norme che servono a delimitare e a dettare un percorso ben preciso, dando al giudice un filo conduttore laddove vi sono controversie di lavoro, questioni delicate da risolvere e laddove vengono indicati alcuni principi ai quali bisogna uniformarsi. al di là di quello che possono essere le soggettive e personali interpretazioni che, come lei sa benissimo, spesso portano a decisioni contrastanti, a decisioni giurisprudenziali, che non vanno verso quel principio della certezza del diritto che dovrebbe essere sempre il traguardo che ciascun legislatore si pone.

anomalo della certificazione. La certificazione, come si dice in parte anche qui, è usata in qualche altro ordinamento per aiutare il giudice ad apprezzare, secondo standard tipici, la qualità tipo contrattuale, ma non per escludere i poteri del giudice. Quindi, confermo che stiamo stravolgendo il sistema in un modo che non ha nessun riscontro in ordinamenti civili. in più si aggiunge che la certificazione verrebbe usata non solo per la qualificazione del contratto - che è l'uso normale che se ne fa anche in altri Paesi - ma anche nell'interpretazione delle clausole contrattuali. Questo sinceramente aggiunge anomalia ad anomalia perché in questo modo si verrebbe ad assolutizzare un carattere del contratto di lavoro come se fosse un qualunque contratto di diritto privato. Sappiamo benissimo, invece, che un contratto di lavoro non è come un contratto di compravendita si inserisce in un quadro normativo ben preciso. Quindi, dire che la certificazione può anche valutare le clausole del contenuto contrattuale a prescindere da qualunque contesto normativo, significa, ancora ancora una volta, non solo alterare le possibilità di correttezza del tipo, ma anche l'equilibrio contrattuale. Quindi, anche questo emendamento è teso a riportare il sistema della certificazione nel suo giusto alveo.

dopo il senatore Benedetti Valentini, avvocato insigne. Come affettuosamente mi ha definito qualche giorno fa il senatore Treu in un simpatico dibattito che abbiamo avuto insieme, sono solo un manovale, nel senso che ho solo l'esperienza, come tanti altri colleghi che hanno fatto sindacato dall'altra parte, di gestire decine e decine di migliaia di dipendenti in giro per il mondo. auspicando il conforto e la benevolenza dei colleghi che sono intervenuti in modo giuslavoristicamente avveduto, chiedo loro di consentirmi una grande sincerità, ai limiti della ruvidezza. Qual è lo scopo dell'articolo 23? Esso, in qualche modo, ci richiama al fatto di aver abbiamo sostenuto la congruità dell'inserimento della riforma del processo del lavoro nel collegato lavoro alla finanziaria. infatti, di fronte a noi un orizzonte nel quale le imprese, soprattutto le piccole e medie, saranno chiamate a poderosi sforzi di ristrutturazione per adeguare strutturalmente le loro capacità produttive al mutato scenario internazionale. Altre imprese, invece, dovranno rimodellare la propria organizzazione per avere un più adeguato riposizionamento competitivo. È allora evidente che potere contare su una riforma profonda del processo del lavoro diventa un vettore

che aveva contestato gli accordi stipulati con le grandi organizzazioni sindacali per gestire ristrutturazioni (pur con tutte le norme protettive per le condizioni individuali),

dei magistrati del lavoro nel perimetro delle relazioni industriali ma addirittura, in qualche misura, di una scarsa considerazione, dovuta spesso al sospetto nei confronti dell'esercizio dell'autonomia delle parti sociali. Noi vogliamo semplicemente dire che, d'ora in avanti, le valutazioni tecniche, organizzative e produttive che le parti sociali o le parti contrattuali assumono a fondamento delle proprie determinazioni

io ho sempre ascoltato con grande attenzione le osservazioni dei colleghi, che questa volta mi onoro di poter chiamare colleghi, Ichino e Treu. In qualche misura, con nessuna superficialità ma con uno straordinario rispetto, ribadisco che crediamo profondamente nel testo prodotto. Non possiamo non considerare come attentamente meditate e degne di profonda riflessione le osservazioni dei colleghi di minoranza. Tuttavia, soltanto la prassi potrà dirci se era giusta la nostra architettura giuridica o se *potiore* sarebbe stata quella proposta, con sincero spirito riformista,

sulla parte relativa al licenziamento state facendo esattamente il contrario di quello che dite di voler fare. Dire che il giudice deve farsi interprete dell'interesse oggettivo dell'impresa è esattamente il contrario rispetto a dire che il giudice deve rispettare la volontà delle parti

fondare la corretta qualificazione. Pertanto, dire che il giudice è vincolato alla volontà delle parti circa la qualificazione del rapporto equivale a dire qualcosa che è destinato a cadere sotto la scure della Corte costituzionale.

siamo perfettamente in grado di produrre gli effetti voluti. Come ha detto il senatore Ichino, noi rischiamo, al di là delle buone intenzioni dei colleghi, di produrre effetti contrastanti. Nel caso del licenziamento questo è chiarissimo. Noi non utilizziamo, come si dovrebbe fare, delle indicazioni collettive e degli standard sociali per indirizzare una valutazione che deve riguardare la legittimità del licenziamento (e non certo

della realtà giuridica di un rapporto di lavoro. Sarebbe come dire che, se le parti dicono che un rapporto di lavoro dipendente è invece autonomo (perché così gli viene),

Temo che non ci rendiamo esattamente conto della portata e della gravità di questa norma. Per favore, riflettiamo e cerchiamo di cambiare questo articolo.

Signora Presidente, l'emendamento 24.300 introduce il concetto della rappresentatività

Signora Presidente, il capogruppo del

«dobbiamo affrontare con cautela questioni molto, molto complesse». una materia che è tra le più complesse che si possano immaginare e considerare, cioè la materia processuale civile. Stiamo intervenendo sul codice di procedura civile. A questo proposito, e proprio in riferimento a questo articolo, il relatore di maggioranza Maurizio Castro, in Commissione ci ha parlato di un processo di "stratificazione normativa virtuosa", vero collega Castro? l'essenza di un codice in un ordinamento civile moderno è esattamente il contrario della stratificazione di norme. Noi qui stiamo manomettendo una una legge, il codice di procedura civile, che dovrebbe essere la quintessenza della semplicità, organicità e sistematicità; interveniamo, invece, con il metodo della stratificazione. Dovrebbe essere principio ovvio di tecnica legislativa quello per cui in un codice - stiamo parlando

Volete un esempio dei pasticci che stiamo facendo? Io chiedo ai relatori se il procedimento di conciliazione di cui parliamo, secondo il vostro intendimento, è un procedimento obbligatorio per entrambe le parti oppure lo è solo per il ricorrente e non per il convenuto. Mi interesserebbe conoscere la vostra opinione al riguardo perché qui state facendo un pasticcio. In una parte della norma In una parte della norma dite che il tentativo è facoltativo ma poi, con il comma 1-*bis*, dite che invece il tentativo di conciliazione è obbligatorio. Una delle due norme è collocata dentro il codice, l'altra è collocata fuori: il comma 1-*bis*,

Voi dite che il giudice deve formulare alle parti una proposta transattiva e poi dite che il giudice dovrà tenere conto, ai fini della sentenza, e quindi dell'esito finale del giudizio, del giustificato motivo di rifiuto dell'ipotesi transattiva formulata. Ma che cosa diavolo può voler dire questo? Facciamo un caso concreto: il lavoratore rivendica 100.000 euro, il giudice fa una proposta transattiva di 50.000 euro il lavoratore o il datore di lavoro rifiuta la proposta transattiva perché evidentemente ritiene di avere ragione prevede che la sentenza gli sarà favorevole. Come può il giudice valutare il giustificato motivo di rifiuto del lavoratore o dell'imprenditore? Questo non ha alcun senso. Se il giudice giudicherà che il lavoratore ha ragione gli darà 100.000 euro. Se riterrà che abbia torto respingerà il ricorso. Ma che senso ha che il giudice debba valutare il giustificato motivo di rifiuto di una proposta transattiva?

probabile causa di impugnazione del lodo? Che ragione c'è di irrigidire con queste regole un istituto che dovrebbe essere il più snello possibile per portare ad una facile soluzione transattiva della vertenza,

il problema dell'arbitrato in Italia sta nel fatto che non è consentito al contratto collettivo di disporre la soluzione arbitrale sui diritti che nascono esclusivamente dal contratto collettivo stesso. Questo è il problema. se noi, come nell'emendamento che abbiamo proposto, dicessimo soltanto questo cioè che il contratto collettivo può disporre la soluzione arbitrale sulle controversie relative a diritti che hanno nel contratto stesso la loro sola fonte, avremmo con questa sola norma deflazionato il contenzioso del lavoro per una metà abbondante. Nella norma che voi ci proponete di approvare facciamo il contrario. Creiamo problemi per l'arbitrato su materia che abbia fonte esclusivamente nell'autonomia collettiva e, viceversa, ampliamo la possibilità di clausola compromissoria a materie disciplinate con legge inderogabile dello Stato; e con questo miniamo alla base il sistema stesso del diritto del lavoro perché un ordinamento in cui la legge detta una norma inderogabile e tuttavia consente alla parte individuale di scegliere un giudice privato che deciderà dell'eventuale controversia in proposito è un ordinamento che si autocondanna alla ineffettività. Quindi, per un verso allargate troppo nella parte sbagliata. Per altro verso, restringete troppo nella parte in cui bisognerebbe invece allargare. È una norma sbagliata. Ma mettiamo pure che io vi stia dicendo delle sciocchezze. Vi sembra che una questione di tale delicatezza, metter mano ad un codice di procedura civile

senza ripetere quanto già detto bene dal collega Ichino, faccio notare che non è che questa materia non era stata considerata. Nella scorsa legislatura abbiamo discusso per mesi un progetto di riforma del processo del lavoro su cui vi era stata una larga convergenza, vi erano state commissioni ministeriali e vi era stata -sottolineo - una convergenza anche di parte dell'opposizione. Adesso mettiamo dentro ad un provvedimento *omnibus* una norma del genere, che non ci sta. Sottolineo due emendamenti significativi: uno vorrebbe recuperare almeno - dato che abbiamo preso questa strada una parte che questa, sì, semplificherebbe le procedure: quella cioè di possibili interventi in materie che hanno carattere di fatto, che riguardano la previdenza e l'assistenza obbligatoria. Tutti i pratici ci dicono che avere una procedura semplice di conciliazione e di accertamento tecnico in queste controversie ridurrebbe la gran parte

qui veramente rischiamo di confondere, altro che di favorire un processo più veloce.

che davvero si misurano due diverse tecniche legislative: è in qualche modo il dibattito che già animò la presentazione della legge Biagi. So benissimo che i colleghi Ichino e Treu siano portatori di una cultura cultura che si ispira al rasoio di Occam e che tenta, secondo noi in maniera forzata, di giungere ad una semplificazione degli istituti. Noi apparteniamo oggettivamente ad una scuola diversa; i risultati che sono stati sinora conseguiti con le nostre tecniche legislative ci confortano nel proseguire, e lo dico con grande semplicità e rispetto. È ben vero che c'è una conciliazione facoltativa e una obbligatoria; quella obbligatoria però è solo quella prevista dall'articolo 80 della legge Biagi. È ben vero che vi sono tre diversi tipi di arbitrato:

Quindi, da questo punto di vista è vero che la nostra è una impostazione di tecnica legislativa che ritiene la complessità un vettore di soluzione adeguata ad una realtà a sua volta *naturaliter* complessa.

costruttivo ai lavori dell'Aula relativamente proprio a questo articolo credo sia necessario segnalare una aporia che è all'interno dell'articolo

412-*quater*, così come scritto, fa riferimento espressamente ad una procedura arbitrale irrituale, ovverosia disciplinata dell'articolo 808*‑ter* del codice di procedura civile. La differenza fondamentale, anzi direi essenziale, con la procedura arbitrale disciplinata da tutti i restanti articoli è che in questo caso non si ha un lodo che ha efficacia di cosa giudicata, quindi equivalente ad una sentenza, bensì si determina un vincolo di natura contrattuale. Fino a qui siamo nel paradigma dell'articolo 808-*ter*. Il problema si pone quando nel testo dell'articolo 412-*quater* successivamente così si afferma: «Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile...». Fino a questo punto siamo ancora nel paradigma civile, perché l'articolo 1372 del codice civile riguarda l'efficacia del contratto e l'articolo 2113 le rinunzie e le transazioni. Il problema si pone subito dopo e si determina in questo caso un'evidente aporia nel sistema prosegue testualmente: «... e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice» - che riguarda l'esecutività dei titoli giudiziari di condanna «a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825». L'articolo 825 del codice di rito è quello in forza del quale le parti, dopo la pronunzia del lodo nell'arbitrato, che dogmaticamente viene definito rituale per distinguerlo da quello irrituale, si rivolgono al giudice per ottenere l'apposizione della formula esecutiva. Orbene, l'articolo 808-*ter,* proprio nell'assoluta consapevolezza del legislatore che un vincolo di natura contrattuale non ha in sé una pronunzia di condanna ma determina soltanto effetti obbligatori (tant'è vero che se non venisse adempiuto si dovrebbe promuovere un giudizio per l'adempimento o l'inadempimento), esclude espressamente il riferimento all'articolo 825, perché nessuna pronunzia avente efficacia contrattuale può essere munita di formula esecutiva. Quindi, si tratta di capire, poiché evidentemente la natura deve essere quella di un provvedimento che ha efficacia di cosa giudicata, che cosa si vuole fare: se è un arbitrato rituale o un arbitrato irrituale. È un dubbio che ripetutamente la Commissione giustizia ha espresso e che è rimasto poi, di fatto, sostanzialmente sospeso in aria.

debbo dire che questa formulazione che fa riferimento alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale mi preoccupa molto nel sistema normale delle relazioni industriali, per vari motivi

Per quanto riguarda la rappresentanze sindacali, una sede analoga non esiste. Non esiste una sede di misurazione di questa consistenza, quindi sulla base di quale valutazione si effettua la misura della consistenza territoriale delle diverse organizzazioni? Abbiamo un criterio nazionale, quello della rappresentatività generale e anche della rappresentatività di queste organizzazioni presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che potrebbe essere uno dei criteri cui si può far riferimento. Voglio sostenere una seconda argomentazione. Attenzione, se ci muoviamo nell'ottica della maggiore rappresentatività territoriale i sistemi di imprese delle aree più forti

sulla relazione industriale, sul costo del lavoro e quindi sulla competitività del sistema che possono essere molto pesanti. In Regioni ad economia più forte abbiamo subito, negli anni, la concorrenza di aree più deboli, che attraverso strumentazioni non di questo tipo, ma analoghe a queste costruivano contratti di lavoro più deboli e venivano nelle aree più forti applicando quei contratti e con quella mano d'opera a fare concorrenza sleale. Vi chiedo di riflettere su tale emendamento, su tale emendamento, perché se l'impianto conciliatorio ha una sua logica per le organizzazioni di imprese, certamente può essere addirittura contrario agli interessi dell'economia territoriale

ma sarebbe un crollo per tutta la comunità, per la città intera. I cantieri Fincantieri devono vivere nell'interesse della città, del tessuto produttivo del Paese, della cantieristica e del tessuto democratico. Ieri, un'interrogazione che chiedeva al ministro Scajola quale iniziativa intendesse prendere per evitare la chiusura e una crisi ulteriore

economico il Governo non si è presentato: questo è gravissimo anche perché erano state intraprese molte iniziative affinché ciò non accadesse. La lotta al degrado e alla criminalità organizzata è anche un'iniziativa contro l'impoverimento economico e la disoccupazione diffusa. In questo momento, presso il Ministero dello sviluppo economico, il sindaco con una rappresentanza dei lavoratori di Fincantieri attende dal Governo una risposta e la convocazione di una data alla quale cominciare cominciare veramente a discutere quali prospettive esistono per Fincantieri. Signora Presidente, le chiedo d'intervenire presso il Governo e di farsi portatore di questo messaggio affinché venga fissata una data per un tavolo al quale effettivamente il Governo partecipi.

la questione da lei evidenziata è sicuramente di straordinaria importanza e rilievo. In questo momento, a quanto mi risulta, è in corso una riunione che attiene esattamente al tema della crisi della cantieristica in Italia, e quindi anche alla vicenda di

mettendole a disposizione 45 milioni di euro finalizzati alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga e che lunedì, a Castellammare di Stabia, ci sarà un incontro con il sindaco e la Regione, al quale io stesso parteciperò, per puntualizzare che all'interno di quelle risorse finanziarie ci sono i fondi relativi alla copertura degli strumenti di tutela per l'indotto Fincantieri, cioè per circa 2.000 lavoratori che altrimenti sono privi di garanzia e di tutela. Ciò non risolve il problema produttivo di Fincantieri, che attiene all'esigenza di recuperare commesse e di trovare continuità dal punto di vista produttivo, tuttavia determina un passo in avanti per garantire un clima più sereno rispetto ai tempi indispensabili per affrontare il tema della ripresa produttiva, che è una questione di dimensioni

distorto delle deposizioni di un pentito, allora è bene ricordare al capogruppo Gasparri che Abu Omar è stato vittima di un sequestro, è stato vittima di un sequestro, che è stato trasportato fuori dall'Italia da agenti dei servizi segreti americani, con la collaborazione di agenti dei servizi segreti italiani, che tutto è stato scoperto attraverso una lunga e faticosa indagine e che Abu Omar non poteva assolutamente aver detto nulla di questo perché si trovava imprigionato in un Paese straniero, dove era stato condotto da chi lo aveva rapito.

un'alta incidenza della camorra, su quanto può incidere negativamente sulla lotta alla criminalità organizzata quello che è avvenuto oggi al Senato. Oggi, infatti, abbiamo

ciò fa molto male a quei cittadini onesti che abitano in luoghi in cui la camorra la fa da padrona.

viene a trovarsi nelle condizioni di dover denunciare o andare semplicemente a deporre davanti ad un magistrato, quando quando in quelle zone lo Stato è stato per molto tempo assente, e lo è anche attualmente, e dà queste manifestazioni. Con queste manifestazioni non si fa la lotta alla camorra, ma la si favorisce!

a fine seduta, dal senatore D'Ambrosio: le respingo al mittente. Voglio ricordare che la vicenda di Abu Omar e dintorni ha comportato un processo ad alcune persone

non compatibile con il suo altissimo e delicatissimo incarico, abbandonandosi ai comizi politico-televisivi che tutti abbiamo visto, esprimendo valutazioni politiche che non gli competono, nello stile tipico della procura di Milano, di cui anche lei, senatore D'Ambrosio, è stato un esponente che ha interpretato in questo modo il suo ruolo. Per quanto riguarda la camorra, noi, in quest'Aula - non so come abbia votato lei - abbiamo inasprito le norme dell'articolo 41-*bis*; abbiamo varato misure severissime per la confisca dei patrimoni delle cosche mafiose e camorriste; abbiamo varato leggi che voi non avete fatto quando siete stati al Governo.

e la violazione del diritto internazionale, dall'altra, per andare contro il terrorismo internazionale tutto hanno a che vedere, tranne che con il garantismo! Se gli argomenti al centro della dichiarazione di voto del senatore Gasparri contro le due mozioni presentate sul caso Cosentino volevano dare prova della grande e piena pratica del garantismo da parte del PdL, tutto viene cancellato in due minuti di replica a fine seduta.